relativamente agli interventi sull'ordine dei lavori e alla disciplina che è stata convenuta

Il Regolamento, come noto ai colleghi, contiene due previsioni distinte tra loro: la prima, contenuta nell'articolo 84, comma 5, che lei ha voluto richiamare, e che riguarda

Ora, se l'oggetto della decisione della Conferenza dei Capigruppo riguarda solo quest'ultima fattispecie, *nulla quaestio* da parte del nostro Gruppo, nel senso che si intende chiarita in questo modo la decisione che lei ci ha comunicato; se invece dovesse investire le altre due fattispecie a cui mi sono riferito (ma credo che ciò non fosse nelle intenzioni di alcuno), allora la questione ovviamente riproposta alla Conferenza dei Capigruppo perché saremmo in presenza di vere e proprie innovazioni regolamentari che andrebbero anche al di là dell'interpretazione della prassi parlamentare

modalità attraverso cui regolare l'andamento dei lavori, in rapporto al fatto che i colleghi dell'allora opposizione utilizzavano questo strumento legittimamente, ma in modo molto esteso. La Presidenza del Senato in quel caso

se ad inizio o a conclusione della seduta. Concludo, signor Presidente, per dire che se l'oggetto della sua comunicazione si riferisce solo alle questioni di minor rilievo, non ci sono problemi e intendiamo acquisita la sua comunicazione; in caso contrario, le chiediamo di promuovere un nuovo pronunciamento della Conferenza dei Capigruppo.

è stato detto nella seduta antimeridiana: la Presidenza, valutata la reale attinenza delle richieste all'andamento dei lavori, si riserva di dare la parola ai richiedenti.

Sono presenti in Aula gli studenti del corso di diritto parlamentare della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova, accompagnati dal professor Paolo Armaroli. Rivolgo ad essi un cordiale saluto.

Onorevoli colleghi, sono stati presentati, poco fa, dal relatore diversi emendamenti al disegno di legge in esame. Come ricordato nella settimana scorsa dal presidente Schifani, gli emendamenti stessi saranno sottoposti al vaglio di ammissibilità ed inviati, per il prescritto parere, alla Commissione bilancio. I Gruppi potranno far pervenire i subemendamenti ai testi in questione entro le ore 20 di questa sera.

in un settore quale quello dell'agricoltura che, per le gravi e diffuse difficoltà in cui versa, richiederebbe un approccio di tipo strutturale. Gli interventi dei senatori del Gruppo del Partito Democratico che mi hanno preceduto ben descrivono l'elenco delle emergenze del settore primario dell'economia del nostro Paese, che mai come oggi potrebbe giocare il ruolo di protagonista nel sostegno alla grave crisi economica e sociale che stiamo attraversando. La consapevolezza è diffusa fra tutti i membri della 9a Commissione del Senato, che a più riprese hanno condiviso punti di analisi e anche di sintesi: prova ne sono alcuni emendamenti da essa approvati in modo unitario. però, non è stata sino ad ora condivisa e sostenuta dalle scelte del Governo. I temi sono, infatti, da diverso tempo in agenda e riguardano interventi che, al pari di quelli oggetto del decreto in discussione, richiederebbero decisioni tempestive. Mi riferisco all'estensione del credito d'imposta a tutte le imprese agricole del Paese, al rafforzamento del sostegno a favore dei consorzi di tutela, all'incentivazione della produzione di biomasse come materie alternative al petrolio ed ai suoi derivati, al ripristino dell'IVA al 10 per cento sull'acquisto di animali vivi, alle agevolazioni in materia contributiva relativa alla previdenza per le aree svantaggiate, al finanziamento dei piani irrigui, alla ristrutturazione del settore della pesca. L'insieme di questi interventi metterebbe in sicurezza il settore, creando le condizioni per affrontare poi una più organica e complessiva ristrutturazione del comparto. Non ho citato un intervento che per urgenza temporale non può attendere oltre e sul quale, proprio per la sua improcrastinabilità, concentrerò il mio intervento. Mi riferisco ai fondi di solidarietà se non si troverà in questo decreto la copertura finanziaria necessaria, metterà in ginocchio sia le aziende incapaci di sostenere gli oneri del rischio derivanti dai nefasti eventi meteorologici, sia le finanze dello Stato il quale sarebbe chiamato ad intervenire con risorse pubbliche alla copertura dei danni, anziché trasferire oneri e rischi a coloro che per oggetto aziendale sarebbero in grado di sostenerli, ossia le compagnie di assicurazione. Il sistema della difesa delle produzioni agricole attraverso l'incentivo dello strumento assicurativo ha infatti dimezzato, dal 2000 ad oggi, le spese pubbliche per il settore, riuscendo a garantire la sopravvivenza delle imprese agricole in caso di calamità. è infatti l'unico comparto economico che, a fronte dell'inflazione in crescita e dell'aumento dei costi di produzione, ha comportato una riduzione della spesa sia per le imprese che per lo Stato. Nella mia regione, l'Emilia Romagna, con un costo di 62 milioni di euro, di cui 48 a carico del Fondo di solidarietà nazionale, sono stati garantiti contro le calamità atmosferiche oltre 945 milioni di produzione a favore di 21.000 aziende che hanno così continuato ad investire. L'allarme degli operatori, non solo emiliano-romagnoli ma dell'intero Paese, è elevatissimo anche perché mancano le risorse che garantiscano la copertura completa della produzione del 2008, anno in cui diverse calamità hanno colpito le colture, provocando danni ingenti sia in termini di quantità, con un perdita media che si aggira intorno al 30 per cento, che di qualità, cosa che si traduce in una diminuzione del valore commerciale della produzione. L'ondata di maltempo dell'ultimo fine settimana sta mettendo in serie difficoltà diverse strutture aziendali, in particolare quelle che Il rischio gelo potrebbe avere effetti disastrosi per molte colture, nella fattispecie quelle in campo aperto. Il vento ha già prodotto danni in serre, stalle e strutture varie; sono stati invasi dalle acque i campi già seminati a cereali e in alcune zone dovrà essere effettuata la risemina. Ancorché la valutazione dei danni da parte del corpo peritale sia ancora in corso, la previsione indica un ammontare di risarcimenti superiore a quanto contabilizzato lo scorso anno. Il Gruppo del Partito Democratico, già in sede di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, aveva individuato tra le priorità del settore il rifinanziamento triennale (corrispondente a circa 200 milioni per anno) del Fondo di solidarietà, ritenendo centrale l'incremento delle risorse necessarie a dare piena attuazione ai meccanismi di gestione del rischio in agricoltura e dando sostenibilità al sistema italiano, che viene indicato come uno dei più avanzati. La Commissione ha votato unanimemente il rifinanziamento annuale: non è quanto chiedevamo, anche se è comunque un risultato; ci impegneremo ancora, affinché possa trovare una copertura, quantomeno triennale, in quanto la sua sostenibilità in un periodo pluriennale è condizione necessaria, sia per assicurare nel tempo il livello di reddito degli imprenditori agricoli, sia per sostenere le scelte per gli investimenti strutturali. Questi ultimi, indispensabili per affrontare il processo di ristrutturazione del settore attraverso processi innovativi, innovativi, restano in capo a coloro che ancora credono nelle potenzialità produttive di reddito dell'agricoltura e vanno quindi incoraggiati. Ciò che si rischia è lo spopolamento delle nostre campagne e non c'è bisogno che qui elenchiamo i grandi danni che questo determinerebbe, non solo in termini economici, ma anche sociali ed ambientali. A fianco a questo, quindi, è necessario mettere in campo tutte le possibili forme di sostegno all'imprenditoria, in particolare giovanile e femminile: interventi, questi, totalmente assenti dal provvedimento

Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, intervengo in discussione generale su un provvedimento che si pone l'obiettivo del rilancio del settore agricolo ed agroalimentare in Italia. un settore nel quale i redditi sono cresciuti del 15 per cento in Europa e diminuiti in Italia di oltre il 3 per cento, con gravi conseguenze produttive ed occupazionali, a costi praticamente triplicati e con redditi sempre più in caduta libera per gli agricoltori italiani, che ormai si collocano in coda tra i Paesi europei. Si divarica la forbice tra prezzi all'origine e prezzi al consumo: per questo, auspichiamo un forte richiamo del *made in Italy* per il settore agricolo ed agroalimentare, che deve essere imperniato sulla centralità dei produttori agricoli e sulla loro capacità di promuovere aggregazioni e filiere economiche in grado di conquistare spazi sui mercati, soprattutto internazionali.

abbiamo bisogno di ammodernare profondamente il settore agricolo ed agroalimentare in termini di competitività delle imprese. Per questi obiettivi abbiamo auspicato misure incisive, a cominciare dalla riduzione dei costi di produzione, agendo sulla leva della fiscalità e della previdenza, nonché sui consumi energetici, con misure finalizzate. Per questi principi, abbiamo puntato sul credito d'imposta su tutto il territorio nazionale, così come avevamo fatto nel precedente Governo. E soprattutto per questo motivo, abbiamo inserito i 200 milioni di euro per il Fondo di solidarietà nazionale (per il rafforzamento e la tutela della competitività dei prodotti a denominazione protetta), il Fondo per il piano irriguo nazionale, le agevolazioni per le aree svantaggiate, per l'acquacoltura per l'acquacoltura e per il settore ittico, per l'imprenditoria femminile e giovanile in un settore, quello agricolo, che rischia una vera e propria senilizzazione. Ecco le proposte del Partito Democratico per rendere più competitivo e produttivo questo settore, perché in un quadro globale stagnante non è possibile pensare di rimettere in moto il Paese senza dare ossigeno al settore agricolo. Troppe le crisi e troppe e fumose le risposte: l'olio d'oliva, che vive una crisi profonda, con costi di produzione sempre più elevati che, insieme alla siccità di quest'anno, rischiano di mettere in ginocchio i nostri produttori, specialmente quelli pugliesi, dove questa produzione occupa il 54 per cento dell'intera superficie La stessa produzione del grano, venduto a costi sempre più bassi a fronte di un prezzo della pasta e del pane che rimane inspiegabilmente troppo alto, specialmente quando importiamo grano di dubbia qualità da Paesi esteri (è di qualche giorno fa la decisione dei coltivatori del Tavoliere di fare lo sciopero della semina, con il risultato di avere pasta italiana, ma non da grano italiano); il parmigiano reggiano, che ha già chiesto sostanziosi aiuti al Governo per continuare a produrre e a difendere il proprio marchio di qualità; la grave crisi del settore vitivinicolo del Tavoliere, quella degli agrumeti di Sicilia, quella dello zucchero, per cui rischiamo di far saltare lo zuccherificio di Termoli e altri due zuccherifici in Italia. La lista della spesa, cari colleghi, è molto lunga e potrei continuare fino all'ora di cena; ci saremmo aspettati quindi una maggiore incisività d'azione da parte del Governo, specialmente per fronteggiare la crisi di mercato delle nostre produzioni e il freno dei consumi dovuto all'aumento prezzi, soprattutto accorciando la filiera. Avremmo voluto vedere più attenzione per fronteggiare l'inadeguatezza infrastrutturale del Mezzogiorno, prima fra tutte la grave crisi idrica di Puglia e Lucania, in quanto sappiamo tutti che l'agricoltura non è solo produzione e fonte di reddito insostituibile, ma garanzia di una corretta gestione del territorio. Le uniche risposte vere sono quelle che abbiamo sostenuto nel precedente Governo, nel solco di quell'attenzione e capacità di ascoltare uno dei settori trainanti della nostra economia. Abbiamo appreso da qualche ora che è stata bocciata ogni forma di agevolazione previdenziale, il fondo di solidarietà, l'imprenditoria giovanile, il fondo ICI: nessun emendamento a sostegno vero dell'agricoltura è stato accolto. Ci dispiace non solo per le sorti di questo settore, ma anche per il paziente lavoro che fino a questa mattina era stato fatto. Debbo pensare che abbiamo solo perso tempo, ne siamo rammaricati ma nel contempo non sorpresi da un Ministro che fa finta di mostrare i muscoli a Bruxelles e non trova il tempo di difendere il suo provvedimento provvedimento in quest'Aula; chieda risposte all'intero comparto, ma anche al Parlamento, sui prezzi, la qualità, i prodotti, l'etichettatura, la sicurezza alimentare. Proprio su quest'ultimo aspetto siamo ancora in attesa di conoscere decisioni in merito alla sorte dell'Agenzia sulla sicurezza alimentare italiana e sulla sua allocazione, decisione già assunta dal Governo precedente e completamente finanziata. Ci auguriamo che il ministro Zaia su tutte queste crisi abbia finalmente il tempo di soffermarsi a guardare al di qua della Linea gotica.

rappresentante del Governo, colleghi senatori presenti in Aula, il settore agroalimentare in Italia è caratterizzato, nelle sue più recenti evoluzioni, da una fortissima attenzione a tutti gli aspetti legati alla qualità, che è estremamente importante perseguire. II settore comprende i prodotti ortofrutticoli, floricoltura, zootecnia e pesca, alimentari, incluso vini e bevande, e circa 70.000 imprese con oltre 450.000 addetti, così come è stato detto negli interventi Il sistema agroindustriale italiano è composto in prevalenza da piccole e medie imprese. La debolezza strutturale è compensata dal fatto che molte aziende italiane offrono prodotti tipici, come è noto, e di elevata qualità, spesso a denominazione di origine controllata, che permettono loro di conquistare tutto un mercato di nicchia, per il quale sono molto appetibili, al riparo della concorrenza dei grandi gruppi industriali, nelle fasce alte del mercato, sia interno che estero. Il 22 per cento del fatturato del settore

il Governo europeo si è impegnato a spingere, sempre di più, le nostre aziende ad avviare nuove relazioni economiche con realtà sia europee che extraeuropee. Ciò ha indotto Ciò ha indotto una serie di innovazioni tecnologiche e un più stretto legame con l'industria e le aziende di servizi; tanto per esemplificare, per le imprese dei settori agroalimentare e prodotti tipici, vendere oltre i confini regionali e nazionali è oggi sempre più possibile anche tramite il "commercio elettronico", sistema che consente di raggiungere immediatamente tutti i possibili acquirenti nel mondo. Tutto questo ha richiesto e richiede continui investimenti. La crisi finanziaria ha portato con sé difficoltà di accesso al credito - passatemi l'espressione - le nostre aziende proiettate sui mercati di tutto il mondo in una palude debitoria tra investimenti fatti o ancora necessari, pagamenti di imposte e introiti non sufficienti a colmare i costi. È un momento molto delicato. La situazione non è migliore per molte delle aziende che hanno nel mercato interno il proprio sbocco naturale: le associazioni dei produttori denunciano il rischio di un crollo della produzione agroalimentare italiana e, specularmente, una vera e propria invasione di prodotti esteri, sulla cui origine e sicurezza alimentare molto spesso c'è da dubitare. Sappiamo che c'è da dubitare ed esempi nel passato recente ne abbiamo avuti; è inutile enunciarli in Il rilancio della competitività del settore agroalimentare italiano all'estero è facilitato dalla legge di conversione del decreto che stiamo discutendo in Aula. a creare migliori condizioni per la partecipazione degli operatori del settore alle dinamiche del mercato e prevede quattro direttrici. La prima sostiene la promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero. Per alcune categorie di imprese viene introdotto un credito d'imposta per gli anni 2008 e 2009 nella misura del 50 per degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi. Tale misura risulta urgente in quanto, dopo un complesso negoziato, la Commissione europea, con decisione C(2008) 668 del 13 febbraio 2008, ha approvato lo schema di decreto attuativo del regime di aiuti; tale disciplina comunitaria non è stata finora recepita per lo scioglimento anticipato della legislatura e conseguentemente occorre rendere operativo l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla norma predetta, al fine di evitare la perdita di risorse finanziarie preziose prefigurate in ambito europeo. L'articolo 1 del decreto, così come definito nella bozza governativa, a mio avviso contiene una limitazione non coerente. Si escludono dal credito d'imposta non tanto le grandi imprese agroalimentari (fatto salvo il caso, per il regime comunitario, degli aiuti di entità minore - aiuti cosiddetti *de minimis* - disciplinati dal regolamento CE 1998/2006),

però rappresentano nel settore il vero *made in Italy*; non solamente nel settore agroalimentare, ma in tutta la produzione del nostro Paese.

e dell'immagine positiva dell'Italia veicolata dai nostri prodotti, dai nostri marchi, dal nostro *made in Italy*. Gli altri punti del decreto riguardano la defiscalizzazione di un contingente di biodiesel, pari a 250.000 tonnellate annue, alcune disposizioni in materia di enti irrigui in Puglia, Lucania e Irpinia e l'adozione del programma SFOP

elencato - che serviranno a dare al sistema agroalimentare una spinta per ripartire nella competizione economica resa oggi difficile anche per l'emergere di nuovi Paesi produttori. Sono certa che un voto favorevole alla legge - ed anche, se possibile, all'emendamento che ho presentato - possa essere più che un segnale di attenzione ai problemi descritti. Un voto favorevole costituirà, infatti, l'occasione di un effettivo momento di rilancio per tante nostre imprese che oggi vedono problematico il proprio futuro. *(Applausi

Sappiamo anche che la manovra finanziaria attualmente all'esame della Commissione bilancio del Senato non solo non interviene con provvedimenti ad ampio respiro nei confronti del comparto agricolo ma, al contrario, prevede tagli strutturali che finiranno per gravare ancor di più su un settore in grave crisi. Oltre a ciò, la disciplina delle quote latte, così come approvata in sede europea, non fornisce garanzie sufficienti, ma anzi rappresenta un'ulteriore zavorra per gli agricoltori.

l'assoggettabilità all'ICI dei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità, siano essi imprese agricole individuali o cooperative agricole. Ho presentato questo emendamento per fugare, una volta per tutte, qualsiasi dubbio di interpretazione legislativa e mantenere così un principio da tempo consolidato. Notoriamente, la Corte di cassazione si era espressa al riguardo con sentenze che hanno stabilito come i fabbricati rurali iscritti nel catasto fabbricati non siano esenti dal pagamento dell'ICI. Con l'accoglimento del mio emendamento si potrebbe dunque chiarire una volta per tutte la succitata questione. A tal riguardo tengo a ricordare che alla Camera dei deputati il Governo, rispondendo ad un'interrogazione del mio collega di partito, onorevole Brugger, si è già espresso a favore di un chiarimento di questa materia promettendo di adoperarsi quanto prima per una soluzione.

In questa fase di acuta crisi economica il settore agricolo non può permettersi tagli indifferenziati e un'ulteriore riduzione di risorse. Il Governo dovrebbe piuttosto abbattere gli oneri burocratici che soffocano questo settore. Auspico che il Governo si mostri sensibile alle questioni da me sollevate, dimostrando di tenere davvero ad un settore portante per la nostra economia, che non può essere abbandonato, specie in un periodo nel quale una vasta crisi economica su scala mondiale sta colpendo tutti, dalle famiglie alle piccole e medie imprese.

disporre per i lavori in modo tale che la 5a Commissione abbia le ore, non i minuti, necessarie per valutare questi emendamenti.

Tale provvedimento, infatti, completa in gran parte il percorso legislativo avviato nel corso della XV legislatura dal Governo Prodi e interrotto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Il decreto‑legge in esame reca, infatti, una serie di misure che già l'allora ministro De Castro aveva deciso di adottare nella prospettiva di rilanciare la competitività del settore agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale. Così anche il provvedimento al nostro esame provvede in tal senso, recando taluni interventi relativi all'adeguamento della normativa agricola nazionale alla disciplina comunitaria, al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo, alle agevolazioni fiscali nel settore delle bioenergie e, infine, provvedimenti che riguardano interventi co‑finanziati dall'Unione europea per gli anni dal 1994 al 1999. Il Governo è dunque intervenuto con il presente decreto-legge al fine di rimediare all'attuale situazione di debolezza del comparto agroalimentare, in particolare con l'articolo 1, che modifica i commi 1088, 1089, 1090 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, relativi al credito d'imposta per la promozione del settore agroalimentare, al fine di consentire alle imprese di sostenere i costi ammessi a incentivo per il 2008, nei termini fissati dalla Commissione europea, e di evitare il rischio di perdere le risorse finanziarie assegnate. La modifica alla legge finanziaria per il 2007 si rende necessaria al fine di adeguare la legislazione vigente, rendendola effettivamente operativa, alla normativa europea, in seguito all'adozione, da parte della Commissione europea, della decisione C(2008) 668 del 13 febbraio 2008, con la quale è stato approvato lo schema di decreto attuativo del regime di aiuti al settore agroalimentare. In sostanza, la nuova disciplina europea, da un lato, consente ad alcune categorie di imprese di beneficiare del credito d'imposta fino al 50 per cento delle spese ammissibili; dall'altro, esclude dal beneficio le grandi imprese agroindustriali - fatta eccezione per il regime *de minimis* - e riduce fortemente le spese realmente ammissibili, escludendo la pubblicità sui prodotti specifici delle singole imprese che, al contrario, la disciplina vigente, introdotta con la finanziaria 2007, ammetteva ai benefici del credito d'imposta. Tale modifica si è resa necessaria in quanto, solamente nel febbraio del 2008, la Commissione europea ha approvato lo schema del decreto attuativo degli aiuti previsti dalla legge n. 296 del 2006. Va ricordato, infatti, che la legge finanziaria 2007 è entrata in vigore il 1° gennaio 2007, mentre lo schema di decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, volto all'attuazione della legge n. 296 del 2006, è stato predisposto e diffuso nel luglio del 2007. Le disposizioni di cui all'articolo 1, che erano già inserite nello schema di decreto legislativo in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, approvato dal precedente Governo il 27 febbraio scorso, prima dello scioglimento anticipato della XV legislatura, devono essere valutate con favore, dal momento che rispondono alle esigenze delle imprese che intendono crescere sui mercati esteri, ampliando le proprie quote di mercato. Inoltre, si tratta di disposizioni innovative, che possono contribuire ad aumentare significativamente la propensione all'*export* del settore agroalimentare italiano. Rispetto al testo della legge finanziaria 2007, va valutato positivamente il fatto che le percentuali del valore degli investimenti, escluse dalla base imponibile del reddito di impresa, siano state unificate ad una sola (50 per cento), mentre precedentemente risultavano diversificate (25, 35 e 50 per cento, a seconda dei casi). L'articolo 2 del decreto-legge al nostro esame proroga al 30 giugno 2009 il termine di utilizzo del contingente di biodiesel defiscalizzato, al fine di evitare l'azzeramento della parte non ancora assegnata nel 2008. Si tratta di una disposizione resa necessaria in quanto le imprese operanti nella filiera devono poter programmare i contingenti di biodiesel con alcuni mesi di anticipo rispetto alla scadenza dell'agevolazione. Si prevede poi che, per gli anni 2008, 2009 e 2010, tale agevolazione fiscale sia attuata dando priorità al biodiesel da filiera, tramite i criteri fissati da un apposito decreto del Ministero dell'economia Per quanto riguarda invece l'articolo 3, con particolare riferimento ai primi tre commi, esso reca una serie di disposizioni nei confronti delle quali noi dell'Italia dei Valori esprimiamo e dobbiamo esprimere una viva contrarietà,

un piano di rientro da trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il decreto stabiliva le procedure amministrative e finanziarie per il «risanamento» dell'Ente. Si prevedeva, inoltre, che, dopo aver proceduto al risanamento finanziario dell'Ente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali avrebbe emanato, d'intesa con le Regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dell'Ente in società per azioni, compartecipata dallo Stato e dalle Regioni interessate. Al fine di concorrere alle esigenze immediate dell'Ente era assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro già nell'anno 2007. Successivamente, con la legge finanziaria del 2008,

mantenendo così in vita il superindebitato e commissariato Ente i cui debiti ammontano ormai a quasi 116 milioni di euro. Mi spiegate con 5 milioni di euro noi che cosa abbiamo realizzato, oltre a dare agli amministratori di quell'Ente 5 milioni da spendere? Lo ripeto: diamo questi soldi alle famiglie degli agricoltori

Gruppo IdV).* L'articolo 4, infine, reca una disposizione che interessa direttamente la pesca cui noi siamo assolutamente favorevoli perché risolve l'emergenza di carattere finanziario e gestionale correlata ai tempi e alle procedure contabili nazionali ed europee, inerenti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione dal 1994 al 1999, valutati in 50 milioni di euro, vengono posti a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Si tratta di una disposizione che oltre a dare conclusione positiva al pregresso amministrativo-finanziario della programmazione per gli anni dal 1994 al 1999, eviterà il blocco degli interventi fra il 2000 e il 2006 del Programma strumento finanziario di orientamento della pesca, sempre a cofinanziamento europeo e in scadenza entro la fine del corrente anno. esprimere apprezzamento per il clima costruttivo in cui si è svolto in Commissione l'esame del provvedimento, trattandosi di materia condivisa sia dalla maggioranza che dall'opposizione, con l'obiettivo del rilancio del settore agroalimentare italiano, finalità questa che deve essere perseguita dal Governo italiano, soprattutto con un impegno in sede comunitaria, per consentire il conseguimento di efficaci norme di tutela e salvaguardia dei prodotti agricoli italiani nonché di rilancio del settore ittico che, come è noto, sta attraversando un momento di forte crisi strutturale, soprattutto in seguito alla crisi energetica in atto.

io sollecito l'approvazione degli emendamenti da noi presentati che sono volti ad incidere in maniera ancora più effettiva a favore delle imprese agricole italiane, nonché a rimuovere dal decreto-legge

Esso è anche necessario, come è stato più volte detto, per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria. Questo provvedimento è atteso da parecchio tempo dal nostro mondo agricolo che sta attraversando un momento di crisi veramente forte. Tale situazione si può considerare solo la punta di un *iceberg* che si è formato, purtroppo, in tanti anni di poco attenta e poco oculata gestione del mondo agricolo, soprattutto per quanto riguarda le trattative fatte in

D'altro canto, la nostra agricoltura merita molta attenzione e merita rispetto. Non dobbiamo, e non possiamo soprattutto, dimenticare i meriti della nostra agricoltura, un'agricoltura che ha permesso al nostro Paese di risollevarsi, soprattutto negli anni immediati dell'ultimo dopoguerra (stiamo parlando dell'inizio degli anni di ripeterlo) un momento di profonda crisi economica. L'agricoltura per il nostro Paese è una vera risorsa primaria e naturale, l'unica vera risorsa primaria e naturale della nostra economia, che si trova, ancora una volta, a svolgere la funzione di trattore e di locomotiva del nostro sistema produttivo. Tale compito, però, non è semplice bensì arduo, visto il momento di non particolare euforia

sta cambiando in maniera radicale la vecchia e sorpassata tendenza dei precedenti Governi. Finalmente, posso affermarlo con piacere, il vento sta spirando in poppa verso la nostra agricoltura.

in tutto il settore agricolo, ma anche nel settore ittico e in svariati altri settori. Egli, però, sta anche recuperando il terreno che abbiamo perso in tutti questi anni di trattative nei confronti degli altri Paesi componenti la Comunità europea. Le lunghe trattative del Ministro a Bruxelles si sono concluse, e qui cito le parole testuali del commissario europeo Fischer Boel, con un lavoro molto pesante a favore dell'agricoltura italiana. I risultati di tale lavoro, bisogna ammetterlo, sono a dir poco eccezionali: abbiamo portato a casa un più 6 per cento sulle quote latte (stiamo parlando di 620.000 tonnellate di latte per un valore di 240 milioni di euro). Questo ci autorizza a parlare di una trattativa storica storica e permetterà a tutto il comparto agricolo di affrontare in maniera più serena e propositiva tutte le questioni del settore lattiero-caseario. Voglio dire che questo provvedimento si staglia anche su altri fronti.

Noi della Lega Nord capiamo che, ancora una volta, bisogna dare una mano e che il Nord deve ancora intervenire nei confronti del Sud. Noi vorremmo, però, con tutta franchezza, che questa fosse l'ultima volta. Vorremmo che i responsabili di quell'Ente facessero un giro dalle nostri parti, in Lombardia, in Veneto in Emilia Romagna, magari copiando e mutuando le gestioni imprenditoriali efficaci ed efficienti dei nostri consorzi, che rappresentano un esempio per tutta l'Italia. le azioni a favore del Fondo di solidarietà per gli incentivi assicurativi. Gli agricoltori ne hanno bisogno per avere un minimo di tranquillità e sicurezza economica nello svolgimento del proprio lavoro. Speriamo anche nella proroga delle agevolazioni previdenziali per i territori montani e per le zone disagiate nello spirito di agevolare ed incentivare il recupero, il presidio ed il controllo di questi territori. positive anche le semplificazioni normative per il trasporto dei rifiuti agricoli. Stiamo parlando di trasporto di modiche quantità fino a un massimo di 30 chili, chiaramente finalizzato al gestore pubblico; provvedimento atteso ormai da anni da tutti i nostri agricoltori, soprattutto dalle aziende medio-piccole. Credo che siamo sulla strada giusta nonostante le non enormi risorse a disposizione da poter investire a favore dell'agricoltura. Oggi i nostri agricoltori hanno sicuramente dalla loro parte una risorsa più: l'ottimismo derivante dall'avere finalmente il Ministro, il Ministero e tutto il Governo che lavorano con loro e insieme a loro, consci delle difficoltà del momento ma con la consapevolezza che l'agricoltura non è più la Cenerentola della nostra economia, ma deve avere ed avrà un ruolo da protagonista nell'economia del nostro Paese.

completa in gran parte il percorso avviato nel corso della XV legislatura ed interrotto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Lo dico anche ai colleghi della Lega:

Al tempo stesso riprende - direi quasi esattamente - il comma 2 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, alimentare e forestale, approvato dal Consiglio dei ministri del Governo Prodi il 27 febbraio 2008. Un'iniziativa che abbiamo giudicato certamente opportuna, anche se ci si poteva spingere oltre per innalzare la capacità competitiva del comparto agroalimentare, soprattutto a fronte della grave crisi mondiale finanziaria ed economica che rischia di avere pesanti ripercussioni sui redditi dei produttori.

più opportune per coprire almeno in parte le esigenze che in vari interventi oggi in Aula abbiamo sentito e che possano dare almeno una risposta parziale ai problemi del settore. Voglio citare solo le più importanti: innanzitutto l'incremento della dotazione di risorse a valere sul Fondo di solidarietà nazionale, necessario per dare piena attuazione ai meccanismi di gestione del rischio in agricoltura e per potenziare il ruolo delle polizze assicurative nazionali; la proroga, per il prossimo triennio 2009-2011, delle agevolazioni in materia di previdenza agricola concesse alle imprese agricole nelle

l'approvazione di tali misure, insieme alle altre proposte emendative presentate dal Gruppo dei senatori del Partito Democratico in Commissione agricoltura (già a partire dalla cosiddetta manovra estiva, dal decreto-legge diventa ancora più determinante nel momento in cui i tagli previsti in finanziaria al settore si trasformeranno - ahimè - in costi maggiori per le imprese, come sarà per la previdenza e le assicurazioni se

Credo - mi rivolgo al ministro Zaia - che al di là delle valutazioni di straordinario successo successo del negoziato di Bruxelles - voglio ricordarle e suggerirgli una qualche prudenza perché in quel negoziato europeo siamo tornati a casa senza nessuna risposta, come lei ha detto, su un settore importante quale è quello del tabacco. Sul tabacco non è stata concessa alcuna proroga per la componente accoppiata degli aiuti e questo comporta la quasi certa chiusura delle aziende nel suo Veneto,

Lei ha parlato di un'ipotesi di luglio, noi aspetteremo, ma non possiamo gridare al successo se un settore così importante non ha avuto alcuna risposta. Vorrei chiosare il collega della Lega sulle quote latte. L'Italia ha avuto un anticipo del 6

Nel testo finale del compromesso si afferma che tale incremento sarà utilizzato per compensare i responsabili del superamento del *plafond* nazionale. Sono certo che lei valuterà con l'attenzione dovuta, perché, accanto a questi signori che hanno splafonato e non hanno rispettato le regole, ci sono più di 40.000 allevatori che hanno rispettato le regole e che hanno anche pagato profumatamente quelle quote che noi oggi rischiamo di dare a chi le regole non le ha rispettate.

all'unanimità anche con l'apporto della minoranza di allora; legge che rappresenta un punto importante, senza dare spazio a illegalità che rischiano di creare seri problemi nella nostra agricoltura.

il provvedimento oggi in discussione riguarda la conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, e rappresenta un'altra importante opportunità per sostenere il sistema agricolo italiano, con interventi fondamentali per rinforzare la competitività e garantire soprattutto la sopravvivenza delle nostre imprese in un periodo di fortissima crisi. L'agricoltura italiana sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia più recente, un'agricoltura sempre più schiacciata dai pesanti oneri economici dei fattori produttivi, dai costi in continua crescita e dall'aumento del divario tra prezzi all'origine e prezzi al consumo. In generale, infatti, mentre i prezzi alla produzione agricola sono diminuiti del 7 per cento lo scorso mese, quelli al consumo continuano ad aumentare generando, da un lato, un calo dei consumi, che riduce le potenzialità produttive delle nostre imprese agricole e, dall'altro, non consentono un'adeguata remunerazione del prodotto agricolo, che in molti casi non copre neanche i costi vivi di produzione, oggetto anch'essi di una crescita fuori controllo. Un quadro complesso che fa emergere e riaffiorare nuovi e vecchi problemi, esigenze che hanno origini lontane e che oggi si sono acutizzate e amplificate a seguito della complessa congiuntura internazionale e che producono un impatto devastante su un sistema ormai da troppo tempo in equilibrio precario. Si deve evitare che da questa crisi l'agricoltura italiana ne venga fuori ulteriormente indebolita, al punto di perdere quella valenza strategica in termini di rinomanza del *made* *in* *Italy* e di veicolo trainante per tutto il Paese. Colleghi, non dimentichiamoci che, nonostante gli occupati nel settore agricolo siano scesi dai circa 8 milioni degli anni Cinquanta al poco più di un milione di oggi, il nostro sistema agricolo ed agroalimentare in genere incide per più del 15 per cento sul prodotto interno lordo nazionale; un dato che fornisce un'importante indicazione sul ruolo che il sistema assume all'interno dell'economia e della società italiana. Un dato che ovviamente è sottostimato in quanto non considera le funzioni plurime che gli imprenditori agricoli svolgono nei territori, ma che fa balzare subito agli occhi il ruolo strategico e primario dell'agricoltura nel nostro Paese. Oggi le nostre imprese agricole, oltre alle storiche problematiche, soffrono le conseguenze della globalizzazione e manifestano difficoltà ad agire in un mercato sempre più esteso e concorrenziale. Nonostante tutto, l'*export* agroalimentare cresce lievemente, soprattutto nei comparti ad elevato valore aggiunto, ma si rafforza l'antagonismo dei nuovi Paesi produttori e spesso i nostri prodotti alimentari pagano pesantemente la sleale concorrenza delle contraffazioni. Si evidenzia quindi la necessità e l'urgenza di una nuova politica agricola e agroalimentare nazionale e comunitaria, un progetto per lo sviluppo ed il rilancio dell'agricoltura, per accrescere le capacità competitive delle imprese agricole, per promuovere e difendere il *made in Italy* alimentare. Dobbiamo evitare che sulle nostre tavole, così come in quelle di tutto il mondo, vengano proposti come prodotti italiani cibi ottenuti da coltivazioni e allevamenti realizzati ben oltre i nostri confini nazionali e con ben altre procedure e norme igienico-sanitarie, come nel caso, ad esempio, del concentrato di pomodoro cinese rilavorato in Italia o delle migliaia di tonnellate di grano duro provenienti dai Paesi extracomunitari e utilizzati per la fabbricazione della pasta. Dobbiamo difendere i nostri prodotti di origine, far uscire dall'anonimato tutte quelle produzioni per le quali oggi non è obbligatorio indicare la provenienza e salvaguardare la fiducia dei consumatori garantendo il monitoraggio e la trasparenza di tutta la filiera alimentare. Colleghi della minoranza, questo decreto‑legge non ha certo l'ambizione e il proposito di intervenire su tutte le problematiche e le criticità che affliggono la nostra agricoltura, il settore agroalimentare, la pesca, l'acquicoltura, sulle quali il Governo è ben al corrente e sta lavorando. Questo decreto-legge rappresenta nello specifico, però, un altro importante tassello di un'azione più complessa e articolata, l'ulteriore conferma dell'impegno che il ministro Zaia e il presidente Berlusconi stanno spendendo per sostenere e rilanciare l'agricoltura italiana a livello nazionale e internazionale. scenari mondiali, la progressiva integrazione del nostro sistema agroalimentare nell'Unione europea, i negoziati internazionali impongono al nostro Governo la scelta di una forte azione di politica estera per la tutela e la promozione del sistema agroalimentare italiano. È di pochi giorni fa, infatti, il grande risultato ottenuto da lei, signor Ministro, a conclusione del negoziato comunitario sullo stato di salute della politica agricola, che vede la nostra agricoltura rafforzata nello scenario europeo e di nuovo protagonista in una trattativa comunitaria. Colleghi, questa per noi è la strada giusta! In quest'ottica è necessario muoversi e in quest'ottica il Governo sta predisponendo tutti i suoi interventi, con strategie che agiscono a breve termine per tamponare le emergenze e con lo studio di azioni di più ampio raggio per mitigare gli effetti dei cambiamenti che riguardano l'agricoltura nel suo complesso. I nostri agricoltori si aspettano non solo interventi immediati ed efficaci, ma anche una politica nuova che non sia né la nostra né la vostra, che non sia né di destra né di sinistra, ma sia il frutto di una strategia di sviluppo che guidi le imprese verso un mercato sempre più complesso e competitivo. Occorre quindi pensare ad un'agricoltura innovata e sempre più presente sui mercati nazionali ed esteri, ad un'agricoltura in grado di contribuire in modo importante alla prevenzione delle calamità naturali, frutto dei mutamenti climatici in atto che stanno cambiando sul campo le regole del gioco e della produzione. Ma occorre pensare anche e soprattutto ad un'agricoltura che si occupi dell'incuria e dell'abbandono del territorio. Occorre ridare valore e dignità all'attività agricola non solo per quanto attiene le tradizionali attività connesse alle produzioni alimentari, ma anche nei riguardi di quelle complementari che vanno dalla protezione ambientale alla produzione di energia. Occorre ragionare oggi in termini di multifunzionalità del sistema agricolo italiano, dove l'impresa agricola diventa il centro di numerose e nuove attività economiche e sociali. Colleghi, non possiamo permettere, così come non lo sta permettendo il Governo, che la nostra agricoltura continui a venire indegnamente considerata la cenerentola della nostra economia. Si tratta di un sistema vitale per il Paese che svolge la funzione di traino per moltissimi settori collaterali, come, ad esempio, l'industria di trasformazione, l'agroindustria, il turismo. C'è bisogno dell'impegno di tutti noi per cambiare il volto e il futuro dell'agricoltura italiana, facendone a pieno titolo un settore primario e sempre più forte della nostra economia e rendendolo sempre più competitivo nei mercati internazionali. bisogna spostare l'asse della competizione dalla quantità alla qualità, dalla competizione sui costi ad una competizione sui territori, dove le nostre imprese, le nostre risorse ed i nostri prodotti, ancorati alle peculiarità territoriali, acquisiscono quel valore aggiunto in grado di farci vincere le sfide internazionali, senza omologarci. Colleghi, come ben sapete, ben sapete, il presidente Berlusconi e, in modo particolare, il Ministro hanno avuto più volte modo di dichiarare, non soltanto in campagna elettorale, che lo stato dell'agricoltura italiana, l'agroalimentare, la qualità, la qualità, la tipicità e la sicurezza dei nostri prodotti sono priorità già inserite nell'agenda di questo Governo. Solo procedendo con le giuste politiche e con i giusti interventi si potrà riguadagnare pian piano in ambito nazionale ed internazionale quella posizione di eccellenza degna della nostra storia e delle nostre tradizioni. Colleghi del Partito Democratico, lo ribadisco, questo non è un decreto-legge che contiene la soluzione finale e definitiva, in grado di rimediare a tutti i mali della nostra agricoltura e del suo grave stato di crisi, ma è un decreto-legge che, come voi avete avuto modo di ribadire anche oggi in quest'Aula, individua una serie di misure fondamentali per il settore agroalimentare. Certo, vista la situazione del sistema agricolo è auspicabile ampliare il raggio di azione e la portata del provvedimento ed è per questo motivo che abbiamo predisposto alcuni emendamenti al testo che sono certo potranno essere da voi condivisi ed appoggiati. Penso, ad esempio, a quello sulla proroga delle agevolazioni previdenziali (per la quale mi appello al Governo), sull'incremento del Fondo di solidarietà o sulla particolare attenzione al settore pesca, giusto per citarne alcuni. Colleghi, e concludo, una cosa è certa: oggi alcuni di voi, del Partito Democratico, si lamentavano di quanto poco c'è in questo provvedimento per l'agricoltura italiana. Io vi ricordo soltanto di quanto poco si parlava di agricoltura fino a poco tempo fa.

e forestali*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, intervengo per sostenere ancora una volta l'importanza strategica del decreto-legge recante misure urgenti per il rilancio competitivo

di un provvedimento che affronta con tempestività ed efficacia i nodi rilevanti cui è esposto il nostro settore agroalimentare. Ho ascoltato con attenzione (al video e di persona) a meno di ricordare che l'agricoltura, la filiera agroalimentare e i nostri territori rurali affrontano in questi mesi una fase estremamente complessa e decisiva per le prospettive future. La crisi economica e finanziaria mondiale esplosa negli ultimi mesi, pur essendo slegata dal settore agricolo, rischia di portare riflessi negativi anche nel nostro comparto per le maggiori difficoltà di accesso al credito, per la sostanziale fragilità dei prodotti spesso non protetti da dazi adeguati, per il rallentamento degli investimenti e, soprattutto, per il calo dei consumi da parte delle famiglie. Un aspetto, quest'ultimo, particolarmente critico per i danni alla domanda internazionale di prodotti dell'agroalimentare *made in Italy* di qualità, che in questi anni ha trainato la costante crescita del nostro *export*,

ho potuto constatare come per troppo tempo al centro dell'attenzione della politica non sia stata l'impresa agricola letta nella sua valenza prevalentemente economica. Così, dopo due anni di prezzi agricoli in rialzo, in questi mesi abbiamo assistito alla rapida inversione di tendenza nelle quotazioni di mercato; in particolare, i cereali (grano duro,

Vi ricordo, tra l'altro, nonostante le polemiche strumentali, che la riunione organizzata per oggi con la filiera dell'olio d'oliva è stata posticipata di comune accordo a giovedì, proprio in virtù dell'impegno del Ministro nella discussione odierna. Anche nel latte le quotazioni sono in rapido calo in tutta Europa per effetto del superamento delle speculazioni internazionali sui derivati e polveri di latte (in Germania il prezzo è calato a 30 centesimi il litro). Questa riduzione dei prezzi agricoli avviene purtroppo con costi di produzione stabili (ricordo che l'urea e l'azoto e quindi tutto quello che è rappresentato dai fertilizzanti è aumentato del 350 per cento negli ultimi sei anni; gli iperfosfati sono aumentati del 30 e pertanto cresce la tensione sui redditi delle nostre imprese. Troppo semplice, forse, ma inevitabile constatare il fallimento delle previsioni su cui l'Europa ha costruito le sue politiche. L'Europa ci ha sempre abituati a ragionare in materia di eccedenze e il risultato di questa sgangherata e disastrosa programmazione oggi ci fa trovare una contabilità negativa; mancano all'appello due milioni di tonnellate di latte rispetto alla programmazione comunitaria, mezzo milione di tonnellate di carne La situazione rimane complicata anche nelle fasi più a valle della filiera. Infatti le difficoltà economiche delle famiglie, la ricerca di prodotti sempre a minor prezzo, nonché la spinta competitiva della distribuzione moderna alimentano tensioni commerciali e purtroppo stimolano i comportamenti di quelle imprese che cercano di muoversi al di fuori delle regole. Per questo oggi diventa importante l'azione del Governo e delle istituzioni locali per il controllo dei prodotti alimentari contro le frodi e le contraffazioni. Abbiamo inaugurato una stagione della tolleranza zero che sta già dando ottimi frutti: ricordo il più grande sequestro della storia di prodotti dell'agroalimentare avvenuto a carico della comunità cinese in quel del porto di Napoli, i sequestri di olio d'oliva, i sequestri in queste ore di grosse partite di vino, i sequestri di burro che comunque non aveva titolo per essere immesso sul mercato e molto altro ancora. Questo è il quadro che dobbiamo affrontare ed è su queste basi che è stata impostata l'azione del Ministero in Italia e in Europa, puntando come mai prima sulla possibilità di dare nuovo slancio a competitività e trasparenza. Il sistema agroalimentare italiano infatti ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo di *leader* in Europa e nei mercati internazionali. Siamo al pari della Francia come agricoltura che produce il maggior valore aggiunto in Europa; abbiamo un modello di produzione orientato più di ogni altro Paese comunitario su prodotti di qualità. Non posso che ricordare i 174 prodotti a denominazione DOP e IGP, il comparto del biologico e tutti i prodotti certificati e non ultimo ricordare che nell'atlante nazionale dei prodotti tipici si possono contare oltre 4.500 prodotti. Quindi, abbiamo grandi potenzialità e non possiamo permetterci il lusso di rimandare la soluzione dei nodi strutturali che frenano le energie di sviluppo di cui sono piene le nostre imprese e i nostri territori. Le imprese devono essere messe in condizione di competere perché solo su queste fondamenta si costruisce la crescita. Competitività e sviluppo sono alla base del negoziato condotto la scorsa settimana a Bruxelles e con il quale l'Italia ha raggiunto risultati straordinari, soprattutto se paragonati a quelli conseguiti nel passato, recente o meno. Prima di tutto il futuro del latte: ne abbiamo parlato in più occasioni in questi giorni e se ne è parlato anche oggi in Aula. Ricordo che il negoziato ci dà la possibilità di avere una disponibilità

raggiunto un altro importante risultato, che è quello di avere oltre 120.000 tonnellate, grazie ad un correttivo sul grasso del latte, da dedicare a nuova produzione. Se a queste 120.000 tonnellate sommiamo le 200.000 frutto delle frutto delle vecchio negoziato (ovvero l'aumento orizzontale del 2 per cento), sappiamo con certezza che abbiamo oltre 320.000 tonnellate da distribuire secondo i criteri della legge n. 119 del 2003 per nuove mungiture.

occorre sottolineare che c'è stato un aumento del 150 per cento del superprelievo nelle prossime annualità, questo ad indicare la direzione della legalità e del rispetto delle regole; ci sarà da parte nostra un impegno a presentare un decreto in Consiglio dei ministri per disporre

considerazioni relative al fatto che spesso non si nota che con questo negoziato abbiamo avuto la possibilità di creare altri due fondi speciali per il latte, uno dei quali all'interno della modulazione che ci ha visto vincitori in un dibattito con il commissario europeo, una modulazione che ci permette oggi di creare, con due nuove possibilità di spesa, pascoli montani e pascoli nelle zone svantaggiate e ci dà la possibilità di investire direttamente sul settore del latte, quindi con il passaggio delle risorse dal primo al secondo pilastro della PAC da dedicarsi ancora indirettamente al mercato.

Questo significa la possibilità di recuperare tutte quelle risorse destinate all'Italia che il nostro Paese non ha utilizzato e che inevitabilmente tornavano all'Europa. Questi sottoutilizzi comunitari ammontano a circa 140 milioni di euro all'anno e verranno impiegati all'interno dell'articolo 68. Dal momento che è stato citato, permettetemi poi di parlare del tabacco, che non era elemento di negoziato, non era nell'ordine dei lavori. Abbiamo insistito in più occasioni perché vogliamo difendere il comparto

e dalla Toscana. Occorre dire che il commissario Fischer Boel si è rifiutato fino all'ultimo istante di discutere di tabacchicoltura; occorre altresì ricordare che abbiamo incontrato i nostri produttori l'ultima volta alle quattro e mezza del mattino per decidere una strategia assieme. Il Ministro non è andato in direzione opposta, ma ha condiviso con i tabacchicoltori una strategia che è quella di non rinunciare alla nostra battaglia in Europa, che è quella di riaprire la battaglia da subito (inizieremo già

Competitività e sviluppo sono anche alla base del decreto-legge in discussione oggi. Con questo provvedimento è iniziato un intervento organico di rilancio del settore attento alle esigenze dei cittadini, delle imprese

Vengono inoltre sbloccati gli incentivi per la produzione di energia elettrica da biomasse in impianti sotto un megawatt. Si tratta di un intervento che permetterà l'avvio operativo di tanti investimenti diffusi di imprese agricole, con effetti benefici anche in termini ambientali (penso ai biogas e al problema dei nitrati). Viene inoltre data attenzione alle imprese con il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale (se ne parlato in più occasioni oggi). Non meno importanti sono le norme per la trasparenza nelle operazioni commerciali delle DOP e delle IGP. completamento, il disegno di legge approvato dal Governo, che sarà sottoposto all'esame del Parlamento, che completa le misure urgenti per il rilancio competitivo del settore primario.

affronta i nodi della trasparenza dei mercati, primo fra tutti il provvedimento sull'etichettatura d'origine dei prodotti agroalimentari, frutto di un accordo strategico con il Ministero dello sviluppo economico, che mette fine ad anni di contrapposizioni tra agricoltura ed industria ed industria alimentare. Questa norma permetterà finalmente di dare certezza ai consumatori e di tutelare il valore delle produzioni agricole.

per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni rese, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge, dopo le parole: "è riconosciuto" siano inserite le seguenti: "nei limiti delle risorse di cui al comma 1090"; che all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge, dopo le parole: "è riconosciuto" siano inserite le seguenti: "nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 Osserva, poi, con riferimento all'articolo 3 del decreto-legge, che appare non conforme alle destinazioni già previste a legislazione vigente il ricorso ad autorizzazioni di spesa di cui viene ridotto l'importo per la copertura di finalità diverse rispetto alle originarie finalizzazioni».

per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.400, 1.401, 1.0.3, 1.0.200 (limitatamente al comma 2), 1.0.4, 1.0.400, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7,

2.0.130. In ordine all'emendamento 1.200 esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che al capoverso Art. 1, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "è riconosciuto" siano inserite le seguenti: "nei limiti delle risorse di cui al comma 1090"; che al capoverso Art. 1, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "è riconosciuto" siano inserite le seguenti: "nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e". Esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte emendative riferite fino all'articolo 2. È rinviata l'espressione del parere sugli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4». riferiti agli articoli 3 e 4». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, a partire dall'articolo 3, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.202, 3.0.200, 3.0.201, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10,

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.0.16, 4.0.18, 4.0.19 e 4.0.22. In ordine alla proposta 4.0.12 il parere è non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, dopo le parole: "al fine di favorire", siano inserite le seguenti: ", nei limiti di tali risorse,". In ordine all'emendamento 4.0.204 il parere è non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che siano inserite, in fine, le seguenti parole: "dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". Esaminati, altresì, gli ulteriori emendamenti, approvati dalla Commissione di merito e trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.0.3 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.0.25 (testo 2), 4.0.37 (testo 2) e 4.0.11 (testo 2). Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti».

un lavoro particolarmente complesso che, tra l'altro, deve tenere conto giustamente anche di quanto disposto, su indicazione del presidente Schifani, nella scorsa settimana relativamente agli emendamenti cosiddetti ultronei.

senatore Andria

il 31 dicembre 2008. La mancata proroga comporterebbe un aumento dei costi della voce lavoro pari al 75 per cento per le imprese agricole nelle regioni ex obiettivo 1 per cento per le imprese agricole nelle aree svantaggiate. Naturalmente, le conseguenze di questa mancata proroga potrebbero essere disastrose per molte aziende già colpite dagli aumenti dei costi di produzione

la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 era solo sul secondo comma.

era il parere unanime della Commissione. Prima avete bocciato la proroga delle agevolazioni previdenziali e adesso abbiamo giocato al ribasso: partendo da 200 milioni di euro per il Fondo di solidarietà siamo arrivati a 70 milioni. Tra l'altro, questa mattina abbiamo a lungo discusso, perché voi sapete che su questo tema è stata presentata un'interrogazione da parte dei senatori del PD, per la copertura dell'anno 2007,

che non soddisfa pienamente, non tanto il Partito Democratico ma gli agricoltori italiani che su questo hanno manifestato nei giorni scorsi. Invito

ci ha oggettivamente precluso la possibilità di passare al voto del secondo comma di questo

cara collega, noi del settore agricolo siamo incappati in questo clima che oggettivamente non è del tutto favorevole alla nostra operatività. Ne prendiamo atto. Del resto, siamo anche consapevoli che successivamente arriveranno altri decreti (vero, onorevole Sottosegretario?), sui quali saremo pronti, incalzanti nei confronti del Ministro perché si possa ottenere per il mondo agricolo e per il mondo della pesca anche quello che non siamo riusciti ad ottenere questa volta. Voglio infine ricordare che, per quanto riguarda il comma 2, c'è la possibilità da parte del Ministero delle politiche agricole e del Governo di poter agire a ristoro almeno parziale dell'interesse degli agricoltori, utilizzando quanto ottenuto con la modulazione in sede comunitaria, grazie all'accordo di Bruxelles della scorsa settimana. Quindi, dal punto di vista pratico stiamo tranquilli e sereni perché per gli agricoltori italiani vi sarà, sia per il 2008 sia per il 2009, un adeguato Fondo di solidarietà.

Per questo emendamento abbiamo rinunciato anche ad una posizione che conteneva una proposta di un recupero di risorse per il triennio. Sappiamo quanto questa proposta sia

la Commissione bilancio lavora sulle risorse e non nel merito. Sarebbe intendimento anche dei commissari tutti della Commissione bilancio dare il più possibile a tutti; purtroppo, il nostro compito è quello di verificare la coerenza tra l'emendamento presentato e le risorse disponibili. D'altra parte, lo facciamo anche in coerenza con il Governo e, nel nostro caso, con il Ministro dell'economia.

pertanto sottolineare, in questi casi in cui tutti i colleghi vorrebbero un maggior numero di risorse, che questo è anche l'intendimento dei singoli commissari di tutta la Commissione bilancio in quanto onorevoli esponenti

signor Presidente, vorrei chiedere quali sono le motivazioni che hanno indotto la Commissione bilancio a rendere improcedibile l'emendamento 1.0.5. Si tratta di una norma d'interpretazione autentica che riguarda l'applicazione dell'ICI sui fabbricati rurali, per i quali l'imposta comunale sugli immobili non è applicabile. Ci sono state una serie di normative successive che hanno richiesto che i fabbricati rurali venissero iscritti al catasto, nulla di questo avrebbe interferito sul requisito dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta, che è legato ai requisiti della ruralità. Quindi, le norme successive non hanno in alcun modo modificato il principio dell'esenzione dei fabbricati rurali dall'ICI, quando questi rispondano ai requisiti richiesti. Ciò è stato ribadito anche da una norma uscita nel 2007, che, mentre modificava le caratteristiche dei requisiti di ruralità, nulla eccepiva circa l'esenzione dall'imposta

sono esenti, a prescindere dal fatto che ad essi sia stata attribuita una rendita catastale e, dall'altro, vi è una sentenza della Cassazione che invece ritiene che questi effetti fiscali non vadano applicati laddove è prevista la determinazione di una rendita catastale.

da una parte, in base alla giurisprudenza, dovrebbero procedere ad accertamenti e richieste di pagamento e, dall'altra, rispettare norme che invece continuano ad affermare che l'elemento soggettivo legato

Quindi, chiedo che anche la maggioranza, che tra l'altro è stata proponente di tale emendamento, che poi noi in sede di Commissione abbiamo fatto nostro e rispetto al quale non riesco a capire perché ci sia una valutazione negativa da parte della Commissione bilancio,

del prossimo decreto che transiterà per quest'Aula. Vorrei avere una rassicurazione perché non potete mettermi in queste condizioni.

tra l'altro molto facilmente e con una disponibilità totale da parte di tutti - e poi vederselo bocciare in modo così brutale. Come si diceva una volta: eccellenza, la esorto ad alzarsi e a darci una risposta positiva,

stiamo valutando l'impatto assieme alla Commissione bilancio.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1 (testo

è stato analizzato poi dal senatore Latronico in Commissione, che ha individuato un solo ente e la relativa copertura. È stato discusso e, a quei sensi, il parere è favorevole.

"3-bis. Il termine del 31 marzo 2009 di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133,

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 200.000 euro per l'anno 2009 l'accantonamento del Ministero dell'interno, e quanto a 50.000 euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Presidente, premetto che, per mia ignoranza, non so cosa sia l'EIPLI, ma è un ente, pubblico o assimilato,

al fine di coprire questo emendamento, qui andiamo a togliere, certo, cifre sostanzialmente irrilevanti; ma, in piena sessione di bilancio, andiamo a ridurre addirittura un fondo di riserva del bilancio a legislazione vigente. Poi, non contenti, nell'ambito di quel fondo di riserva e, più in generale, per il 2009, tocchiamo

quale sia e cosa faccia questo ente), ma vi pare il caso, colleghi della maggioranza, lo chiedo anche al relatore e al Governo, di dare pareri favorevoli su emendamenti con questi caratteri? Non vi sembra ragionevole che, se il decreto è tale per le misure urgenti che contiene, che riguardano lo sviluppo, in questo caso nel settore dell'agricoltura, ci si dovrebbe contenere in modo tale da evitare "marchette"

voglio qui precisare che l'Ente irrigazione viene destinato ad esercitare un'attività che rientra nelle competenze delle Regioni interessate e che sicuramente può essere sciolto com'era stato previsto da una legge dello Stato e come era stato definito attraverso un accordo delle due Regioni interessate. Ritengo quindi che questo emendamento non solo sottragga risorse ad altri capitoli importanti, come già sottolineato dal senatore Morando, ma alimenti una attività della quale lo Stato può tranquillamente fare a meno. Approfitto della parola per segnalare la mia contrarietà all'emendamento 3.203, perché, mentre da una parte si vuole far sopravvivere una superfetazione di carattere statale, dall'altra si vuole imporre alle Regioni e - cosa ancor più grave - ai soggetti utilizzatori, cioè all'agricoltura, delle tariffe all'ingrosso costruite non già su un progetto industriale orientato all'efficacia e all'efficienza, bensì per alimentare gli sprechi e le disfunzioni che si sono determinate sin qui. Per questo motivo,

per portare quell'opera in giro per il mondo: quindi, di marchette abbiamo avuto un grande esempio. In questo caso non si tratta assolutamente di quel comportamento farneticante a cui si è assistito allora in quest'Aula, che determinò la caduta di quella maggioranza, ma si tratta di ben altro: si tratta di mantenere in vita un ente

integerrima trasparenza abbiamo avuto grande esempio in quest'Aula, anche in occasione dell'approvazione di quegli emendamenti da cui egli si dissociò. Pertanto, ho grande dispiacere per quello che sta avvenendo e chiederei

Presidente, intervengo a sostegno dell'emendamento 3.0.90, che prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro a sostegno del Piano irriguo nazionale.

che possiamo sostenere uno stanziamento per un ente irriguo e non sostenere il finanziamento per migliorare la nostra rete infrastrutturale, che riguarda ovviamente il fondo irriguo nazionale. Richiamo alla coerenza degli stessi colleghi che hanno votato gli emendamenti precedenti, soprattutto ai firmatari delle Regioni Puglia e Lucania. Debbo dire anche che, nonostante l'impegno della stessa Commissione, il Governo, tra l'altro smentendo sia la Commissione che la stessa maggioranza, ha ritenuto di decidere difformemente. Ritengo che dobbiamo sostenere il

Voglio però notare che la Commissione bilancio è stata particolarmente scrupolosa, così come nelle altre occasioni, nei confronti degli emendamenti che sono stati presentati, o da noi o, il più delle volte, comunemente, con uno sforzo congiunto, da parte di maggioranza e opposizione.

che dalle parole si passi rapidamente ai fatti e che quindi il rappresentante del Governo possa confermarci che nella prospettiva anche di una proposta di legge di

Termino, signor Presidente, con una piccola nota d'ambiente relativamente a quanto lei cortesemente mi ha detto quando sono stato apostrofato, insieme agli altri colleghi,

dare dei "marchettari" ad altri colleghi, caro Presidente, non è assolutamente tollerabile. Non è l'espressione di un parere, non è l'espressione di una valutazione, non è l'espressione di alcunché. È semplicemente un'offesa, almeno

agricole che da sempre combattono con la burocrazia. Con l'approvazione di questo emendamento faremmo sicuramente un passo in avanti perché razionalizzeremmo gli impegni delle aziende agricole, ma soprattutto lavoreremmo a favore dell'ecologia, combattendo l'abbandono dei rifiuti.

1985, n. 124. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

relativo alla previdenza, si tratterebbe di un emendamento di complessità straordinaria che merita il tempo necessario. È notorio che io sui contributi agricoli unificati ho condotto battaglie per anni. Sono profondamente convinto che un